Desidero puntualizzare, in primo luogo, in relazione alla possibile presenza di elementi in uranio impoverito nel velivolo C-130J matricola militare 62176 - numero di serie del costruttore 5497 coinvolto nell'incidente del 23 novembre 2009, che il velivolo in questione è di versione 382U (versione corta) e, pur avendo il *serial number* superiore a 5536, non ha equilibratori con elementi in uranio impoverito. Chiarito questo aspetto, osservo che la documentazione tecnica richiamata nell'interrogazione - ovvero, il *Technical Order* (T.O.) 00-105e-9, di cui poi fornirò copia all'interrogante, costituisce il manuale tecnico d'informazione contenente le procedure generali da condurre in caso di emergenza o di incidente, elaborato da *Air Force Civil Engineer Support Agency* (AFCESA) e recepito dai Paesi aderenti alla NATO quale procedura standard per gli interventi in caso d'incidente attraverso lo *Standardization Agreement* I contenuti del documento citato sono finalizzati anche ad indicare parte degli elementi tecnici di dettaglio di ogni tipologia di aeromobile, così da facilitare, in situazioni di necessità, le operazioni delle squadre d'intervento.

riporta, invece, al paragrafo 1-2.5.8. una tabella di relazione tra le versioni del velivolo C-130J acquisite dall'aeronautica militare, i numeri di serie della ditta e le matricole dell'aeronautica militare: da questa tabella si evince, per l'appunto, che il velivolo incidentato è di versione corta.

un paragrafo intitolato "Contrappesi in uranio'', dove viene specificato che solo sui velivoli di versione 382V (versione lunga) i contrappesi interni delle superfici mobili dei piani di coda possono essere in uranio impoverito.

cinque velivoli, in data 8 dicembre 2008, è stato firmato con Lockheed Martin Aeronautics Company un contratto che prevede la sostituzione di detti particolari con elementi in tungsteno sinterizzato e lo smaltimento delle parti in uranio impoverito, con trasporto negli USA, a cura e onere della ditta stessa. Quanto, in ultimo, alle procedure da adottare a seguito di incidenti in cui siano coinvolti velivoli dell'aeronautica militare, voglio rassicurare i senatori interroganti sulla circostanza che è prassi dei reparti di volo di Forza armata fornire agli enti ed agli organi locali interessati copia dei propri piani di intervento. Ciò, proprio al fine di gestire in maniera coordinata le eventuali attività di soccorso,

contrappesi in uranio impoverito fino al numero di serie 5536. C'è poi la distinzione tra il modello lungo e quello corto che, in realtà, è abbastanza informale e di cui non è facilissimo trovare asseverazione sicura perché,

che potremo ove necessario produrre, ci dice che l'ufficio stampa della Lockheed Martin ha fornito, per iscritto, il numero di serie del C-130J precipitato. Esso è purtroppo il 5437, 5437, un numero che precede di gran lunga il 5536, cioè il numero a partire dal quale su alcuni di questi modelli non sarebbe stato caricato l'uranio impoverito, ma il tungsteno.

Resta, sotto questo profilo, un dubbio stringente sul fatto che su quel velivolo potessero trovarsi 64 chili di contrappesi di uranio impoverito nelle ali che sono montate anche sugli altri modelli.

in un formulario specifico - che la massima esposizione all'uranio impoverito, in caso di evento catastrofico, riguarda i vigili del fuoco impegnati nello spegnimento dell'incendio e il personale dedicato a ripulire il sito dell'incidente.

i vigili del fuoco sono entrati in contatto con questa materia pericolosa, noi, a tutt'oggi, ancora non possiamo saperlo; peggio ancora, il comandante dei vigili del fuoco, il funzionario Paolo Gavina, riferisce che per spegnere le fiamme tra i rottami del C-130J C-130J sono stati utilizzati solo acqua e schiumogeni e che i vigili del fuoco non erano a conoscenza della possibile presenza di uranio impoverito. Penso che in questa circostanza un minimo di precauzione, secondo il principio di cautela, si sarebbe dovuto prendere: non si poteva mandare gli uomini a spegnere l'incendio senza senza dar loro un minimo di preparazione in merito. Concludo dicendo che la questione dell'uranio impoverito è purtroppo allargata a ulteriori vicende, su cui sarò costretto a intervenire con altre interrogazioni. La senatrice Franca Rame, che nella legislatura precedente si è occupata a lungo

delle richieste di singole famiglie, una quantità di barocche ostruzioni che rende impossibile, soprattutto per famiglie non abbienti, che non hanno la possibilità di rivolgersi ad avvocati di grido, il raggiungimento dell'obiettivo. perciò che la risposta del Governo non mi soddisfa e che noi siamo pronti a proseguire questa indagine e a fornire nel prossimo futuro dettagli che consideriamo importanti per la conoscenza delle Assemblee rappresentative, perché non possiamo tacere

Con riferimento all'interrogazione dei senatori Vita e Marcucci, con la quale chiedono di conoscere le motivazioni dell'esclusione della Fondazione Giuseppe Di Vittorio dai finanziamenti statali, faccio presente quanto segue. Le domande di ammissione dei vari istituti culturali al contributo ordinario dello Stato per il triennio 2009-2011 sono state valutate da una commissione istituita appositamente con decreto del direttore generale per le biblioteche e gli istituti culturali del 28 ottobre 2009. Quest'ultima ha svolto un esame comparativo delle istanze pervenute, utilizzando quale parametro di valutazione i criteri puntualmente disciplinati dalla legge

della legge n. 534 del 1996. In particolare, è stata riscontrata la carenza del "rilevante patrimonio bibliografico, archivistico, museale [...] pubblicamente fruibile in forma continuativa" e la mancanza della "catalogazione e applicazioni informatiche finalizzate alla costruzione di basi di dati e di immagini", requisiti che la legge citata pone come condizione essenziale per ottenere il contributo.

Tuttavia, onorevole Giro, più che dichiararmi insoddisfatto (come nella retorica consueta si usa dire, a seconda che si sia più, meno, tanto, appena appena o magari persino un po' soddisfatti), la mia replica - non so se ciò è usuale in quest'Aula - è di incomprensione della risposta. Intanto c'è una non coincidenza temporale (mi permetta, signor Sottosegretario, forse non ho colto bene le sue parole): l'interrogazione è del 20 ottobre 2009, ha fatto riferimento ad un qualche atto del 28 ottobre 2009. Dunque, c'è una discrasia: l'interrogazione è precedente. Peraltro, come si può immaginare, l'interrogazione in genere non è improvvisata al momento; ha almeno qualche ora di istruttoria (incontri, conoscenza delle questioni e così via). Vorrei pertanto invitare lei, come rappresentante del Governo e il suo Ministero

parlo di personalità che hanno avuto a che fare con il mondo politico, ad esempio).

con riferimento alle richieste di informazione degli onorevoli interroganti sui finanziamenti ai progetti sull'accessibilità delle persone disabili alle novità librarie, si fa presente quanto segue. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, datato 18 dicembre 2007, a firma dell'allora ministro Rutelli, relativo all'attribuzione dei finanziamenti in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti, veniva fissato il 7 maggio 2008 quale data ultima di presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti da parte delle case editrici. A tale scadenza sono pervenute 13 istanze progetto. Successivamente, con decreto ministeriale datato 16 settembre 2008, il ministro Bondi ha istituito una commissione con lo specifico compito di valutare i progetti presentati, secondo quanto indicato dall'articolo 4 del citato decreto ministeriale del 18 dicembre 2007. La commissione si è insediata presso il centro per il libro e la lettura il 22 ottobre 2008 ma, a causa delle dimissioni di alcuni componenti nel periodo compreso tra i mesi di febbraio e marzo del 2009, la sua composizione è stata modificata con un ulteriore decreto ministeriale, datato 8 maggio 2009. Si rappresenta inoltre che nel corso di svolgimento dei lavori è stata sollevata, nella riunione del 7 luglio 2009,

possibilità di erogare contributi ordinari annuali alle istituzioni culturali non inserite nella tabella. Fa presente che è imminente la conclusione del procedimento.

nel dicembre del 2009 non abbiamo capito se ha concluso o meno i suoi lavori per esaminare 13 istanze di progetto,

quindi senza alcun problema di ordine finanziario. Nel frattempo abbiamo adottato alcuni provvedimenti legislativi

appositamente predisposti perché con la strumentazione di lettura egli riesca, o in forma audio o in forma tattile, ad accedere ai testi. Non c'è neanche bisogno di sottolineare al Sottosegretario ed ai colleghi qui presenti che questo rappresenta la vita per un non vedente:

cercare di dare un aiuto a queste persone sfortunate. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, le

progetti sono stati finanziati ed a che punto sono. Soprattutto mi sarei aspettato dalla sensibilità del Sottosegretario anche una

consente ai non vedenti di sottoporre a scansione un libro per ottenerne il *file*, ma non permette loro di scambiare quel *file* con altri disabili.

culturali*. In merito a quanto rappresentato dalle onorevoli senatrici interroganti circa le difficoltà finanziarie delle istituzioni scolastiche, vorrei in primo luogo fare presente che, diversamente da quanto affermato nell'interrogazione, la sofferenza finanziaria delle scuole per l'anno 2008 è stata determinata dall'applicazione della cosiddetta norma di salvaguardia, contenuta all'articolo 1, comma 621, lettera *b)*, della legge finanziaria 2007, varata dalla precedente amministrazione. Questa disposizione ha, infatti, previsto interventi compensativi, previo decremento degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione relativi ad altre voci di spesa diverse da quelle di personale, da operare a fronte dell'eventuale mancato raggiungimento delle economie da conseguire a seguito del processo di razionalizzazione del personale docente e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, previsto nell'articolo 1, comma 620, della medesima legge finanziaria 2007. Poiché per l'anno scolastico 2007-2008 dette economie non sono state realizzate, a seguito della rimodulazione delle stesse, operata dall'articolo 2, comma 412, della legge finanziaria 2008, si è proceduto, per l'anno 2008, ad una riduzione di 560 milioni di euro degli stanziamenti di bilancio

appena insediato, mediante l'integrazione di 200 milioni di euro della stanziamento del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, disposta con l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, Le criticità finanziarie rappresentate sono dunque da porre in relazione all'applicazione della suddetta norma di salvaguardia, introdotta nella precedente legislatura, e derivano dalla decisione della precedente amministrazione di non procedere alla prevista razionalizzazione degli organici del personale della scuola. Quanto all'ultima *tranche* degli stanziamenti previsti per il 2008, di cui nell'interrogazione si lamenta il mancato invio, si assicura che la stessa è stata già regolarmente accreditata alle scuole. Risulta infatti che sono stati integralmente erogati a favore delle istituzioni scolastiche tutti gli stanziamenti del 2007 e del 2008, sia per quanto riguarda le spese di personale che per le spese di funzionamento. Per l'anno 2009 gli stanziamenti relativi alle spese di funzionamento delle scuole ammontano ad 675.896.750 euro contro contro 538.221.356 euro del 2008, con un incremento quindi di 137.675.394 euro, mentre per le spese relative alle supplenze brevi lo stanziamento per il medesimo anno

267.752.080 euro. Per il 2010, il Ministero continuerà a monitorare attentamente le necessità finanziarie per il funzionamento delle scuole ed interverrà, se del caso, anche in sede di assestamento del bilancio, come già fatto nell'esercizio 2009, assegnando per il funzionamento delle istituzioni scolastiche risorse aggiuntive

i dirigenti scolastici, con regolare bollettino, stanno chiedendo soldi alle famiglie per la normale gestione. Ciò non era mai successo;

che non c'è più margine orario per coprire le supplenze brevi con il personale, che prima aveva un minimo di "gioco". Alla faccia dell'autonomia scolastica, che dovrebbe essere garantita dalla Costituzione, nonché dal Governo più federalista della storia repubblicana!

la mobilità dei docenti", come è noto al senatore interrogante, è il decreto ministeriale n. 45 del 23 settembre 2009, con il quale sono stati fissati i criteri di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario. L'articolo 5 del decreto medesimo prevede "interventi per favorire la mobilità del personale docente e ricercatore" verso le "facoltà nelle quali il rapporto tra studenti iscritti...e docenti di ruolo sia superiore al valore mediano nazionale di tale rapporto nelle facoltà dello stesso gruppo": nel caso specifico il valore è stato fissato in 20,76 allo scopo dì favorire nell'ambito del gruppo delle facoltà di farmacia, il riequilibrio tra facoltà con maggiore e minore docenza. Inoltre, l'articolo 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dispone che, a decorrere dall'anno 2006, le Università, anche al fine di perseguire obiettivi di efficacia e qualità dei servizi offerti, entro il 30 giugno dì ogni anno adottano, con decreto, programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo, sentiti la Conferenza dei rettori, il Consiglio nazionale universitario ed il Consiglio nazionale degli studenti universitari, tenendo anche conto delle risorse acquisite autonomamente. I suddetti programmi individuano in particolare i corsi di studio da istituire ed attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere. Pertanto, sono le stesse università a decidere, compatibilmente con le risorse disponibili, sempre nell'ambito della suddetta programmazione triennale ed in piena autonomia, il fabbisogno di personale docente da reclutare per il settore scientifico disciplinare e, conseguentemente per le singole facoltà.

prendo atto della sua risposta, della quale mi dichiaro soddisfatto, pur evidenziando che l'impegno del Governo

per la facoltà di farmacia verso quel rapporto mediano che segna il punto di riferimento, il parametro di tutte le facoltà tecnico-scientifiche. In quell'ambito il rapporto mediano viene individuato intorno a 7,

di figure professionali che hanno, anche a seguito di recenti provvedimenti normativi, una funzione particolarmente rilevante nella garanzia di accesso ai servizi socio-sanitari anche di tipo territoriale, oltre a profili professionali legati all'attività di ricerca di un settore straordinariamente importante, che rappresenta un volano dell'economia. Quando si parla di ricerca farmaceutica si fa riferimento ad un settore che non soltanto dà risposte importanti alla crescente crescente domanda di salute, con riferimento anche a vecchie e nuove patologie, ma che assume un rilievo anche sotto il profilo del prodotto interno lordo, per

che il Governo per suo autorevole tramite mi fa giungere, vi sia progressivamente il recupero di questo *gap*, che non può essere tollerato più a lungo